Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Desidero anzitutto ringraziare i Presidenti delle Commissioni, i rappresentanti del Governo che hanno partecipato in questi giorni alle sedute di Commissione, il correlatore, collega Laus, e tutti i componenti delle Commissioni riunite per il lungo lavoro svolto per migliorare il testo, cercando di dare una risposta alle problematiche emerse nel corso del dibattito. Andando subito nel dettaglio del contenuto del provvedimento, rilevo che l'articolo 1 rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, rimettendo i termini dei contribuenti che hanno usufruito di tali benefici con riferimento alle rate dovute nel 2020 e nel 2021. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite, questi pagamenti che ho citato (per intenderci rottamazione-*ter* intenderci e saldo e stralcio) sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Sul tema evidenzio che accogliamo con favore l'impegno del Governo a prorogare e dilazionare ulteriormente tale scadenza (mi riferisco sempre alla rottamazione-*ter* e al saldo e stralcio) nel corso del 2022. L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, portandolo per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da sessanta Questo termine è stato portato a centottanta giorni da un emendamento condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, quindi le cartelle notificate a decorrere dal 1° settembre 2021 avranno scadenza di pagamento a centottanta giorni e non a sessanta, come prevede il termine ordinario. Il successivo articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista tra l'altro una decadenza molto lunga del beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di 18 anziché di 10 rate anche non consecutive. È stato approvato un emendamento proposto da noi redattori che rimette nei termini le rate degli avvisi bonari che erano state sospese da marzo a maggio 2020 e che avevano termine ultimo di versamento il 16 settembre e il 16 dicembre 2020. Sono stati approvati altresì emendamenti recanti semplificazioni amministrative, disposizioni che consentono agli operatori sanitari (quindi farmacie, ottici, eccetera) di continuare ancora per un anno ad effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle spese sanitarie (ad esempio i medicinali)

per l'emanazione delle regole tecniche volte a definire le caratteristiche di sistemi evoluti di incasso mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; l'estensione al 2022 del divieto di emettere fatture elettroniche tramite sistema di interscambio, sempre per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche; la previsione di un obbligo, per gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i predetti strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA Spa, i dati che identificano univocamente gli strumenti utilizzati dall'esercente, nonché l'importo complessivo giornaliero dei pagamenti elettronici eseguiti mediante tali strumenti. Al fine di arginare, seppure in parte marginale, la crisi di liquidità causata dalla lunga chiusura degli impianti sportivi, è stata introdotta una disposizione che prevede il rinvio di tutti i versamenti dovuti a titolo di imposte dirette e indirette in scadenza dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021. L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, disciplina la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione di premi della lotteria dei corrispettivi. Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente. I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di quei soggetti che li hanno utilizzati indebitamente. Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite è stato approvato l'emendamento che sopprime il comma 14 che, modificando l'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, dispone che i revisori legali vengano fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e quindi all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997. di importanza anche l'approvazione dell'emendamento che risolve la problematica relativa ai criteri di individuazione della platea beneficiaria del fondo che si rivolge alle attività di *bed and breakfast* a gestione familiare e non avente carattere imprenditoriale, che pertanto non necessitano di iscrizione presso la Camera di commercio. È stato altresì approvato un emendamento che risolve la problematica del canone unico patrimoniale, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale realizzata con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali, che prevedono che il canone sia corrisposto dal titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo di materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione medesima. L'articolo 6 sostituisce alla disciplina del *patent* *box* che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni materiali, giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. In relazione alle problematiche che sono emerse proprio sull'articolo 6 e, quindi sulla nuova disciplina del *patent* *box*, nel corso del confronto parlamentare, il Governo ha comunque rassicurato che la questione sarà risolta in sede di legge di bilancio. L'articolo 7, signor Presidente, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro la dotazione del fondo per la concessione sia dei contributi Ecobonus per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissione superiori nonché per gli autoveicoli commerciali speciali e usati. In sede di esame del provvedimento è stato approvato il rifinanziamento del fondo automotive in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti, il cosiddetto retrofit, al fine di trasferire al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le competenze relative alla gestione dei contributi.

Ringrazio anche per avermi concesso di esporre la relazione.

collega Fenu. Ringrazio i rappresentanti del Governo, la presidente della Commissione lavoro, collega Matrisciano, e il presidente della Commissione finanze D'Alfonso. Non sono dei ringraziamenti formali, ma di sostanza. Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e un ringraziamento particolare alla preziosa collaborazione che hanno voluto e saputo dare i colleghi delle opposizioni. Riguardo alle norme del presente decreto relative all'area lavoristica o sociale, si segnala, in primo luogo, l'articolo 8. Il comma 1 di tale articolo modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale l'applicazione - a determinate condizioni - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero. Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale - tutela che, secondo l'interpretazione seguita, non poteva, a normativa vigente, trovare applicazione, per i lavoratori dipendenti privati, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020

a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020. Si stabilisce, inoltre, l'introduzione di uno stanziamento pari a 188,3 milioni per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento a determinate condizioni di un rimborso forfettario relativo sia al 2020, che al 2021 in favore dei datori di lavoro privati per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS. Si stabilisce altresì l'esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzione previdenziale presso l'INPS. In particolare, le fattispecie in oggetto concernono, in alternativa tra i due genitori e con riferimento a un figlio minore di anni quattordici e convivente, per i periodi relativi al medesimo periodo di sospensione dell'attività didattico-educativa in presenza di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Si prescinde dall'età del figlio nonché dai requisiti della convivenza e della fruizione in via alternativa all'altro genitore qualora le fattispecie suddette riguardino un figlio in condizioni di disabilità grave. Inoltre, per la medesima ipotesi di figlio in condizioni di disabilità grave si riconosce il diritto in esame anche per il caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. L'astensione può essere effettuata in forma giornaliera od oraria. La relativa indennità è riconosciuta dall'INPS, ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro. Per i lavoratori dipendenti l'indennità è pari al 50 per cento della retribuzione che sarebbe spettata, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono l'inserimento di un articolo 9-*bis*, ai fini della revisione e dell'attuazione della recente norma che ha istituito un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento. Il comma 1 dell'articolo 10 prevede che, per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, il trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso anche per un periodo successivo alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria; nel testo proposto dall'emendamento approvato dalle Commissioni riunite, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 1'ambito di applicazione di una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro; in base alla disposizione oggetto di proroga, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo al fine di consentire la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, del quale vengono integrate le finalità, Con tale articolo aggiuntivo, inoltre, in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono riformulate le disposizioni istitutive del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. medesimo. Una importante scelta di giustizia sociale che rappresenta in modo concreto una risposta a un'ingiustizia denunciata da molte famiglie e associazioni. Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite, si estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite, si prevedono un complesso di benefici in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico e dei relativi datori di lavoro nonché alcune misure in favore delle start-up a vocazione sociale. Si tratta di una modifica che porta anche

che assumono, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico nella misura di due terzi del personale. Ciò consentirà la nascita di realtà che hanno come obiettivo l'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche. Il comma 1 dell'articolo 13 - insieme con l'Allegato 1 - reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro; le Commissioni riunite propongono peraltro una serie di ulteriori integrazioni specifiche nonché l'inserimento di un articolo aggiuntivo relativo alla sicurezza sul lavoro nel settore scolastico. Tra le modifiche vorrei segnalarne una a cui tengo molto, che sanziona in modo chiaro l'abuso e l'uso improprio del lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine e che prevede che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, alfine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Mi auguro che ciò rappresenti finalmente un deterrente per l'abuso di queste forme scorrette di "lavoro". di "lavoro". Inoltre, è stato approvato un emendamento che definisce normativamente la figura del preposto. L'introduzione del rafforzamento della figura del preposto è il primo passo per garantire un controllo interno che si affianca ai controlli esterni dell'ispettorato nazionale del lavoro che, con questo decreto, esce potenziato per competenze e per numero di addetti. un altro emendamento consente poi ai lavoratori, alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati di svolgere una formazione specifica in materia di sicurezza per far sì che tutte le persone che avranno l'incarico di occuparsi

In questi giorni le Commissioni competenti hanno lavorato moltissime ore, ma purtroppo, troppo spesso, dai banchi del Governo ai partiti è stato risposto: noi diamo una visione laica. Per i partiti non esiste una visione laica, ma esiste una visione sentimentale della politica, perché vogliamo tutelare i cittadini, al di là dei regolamenti amministrativi vincolanti, di chi opera solo sotto l'aspetto tecnocratico e burocratico. La politica deve dare delle risposte e per questa ragione abbiamo presentato emendamenti, condivisi

Troppo spesso la tecnocrazia dimentica che i cittadini soffrono se non hanno sicurezze e certezze e per questo vogliamo sconfiggere la tecnocrazia, riportando il sentimento nella politica e nel Governo. È questa la lotta dei dei parlamentari della Lega e quindi ringrazio i senatori Augussori e Ripamonti, che in questi giorni, insieme a tutti gli altri colleghi, si sono battuti per difendere i lavoratori fragili. Il senatore Ripamonti, ad esempio, con un emendamento tutelare i cittadini di Savona, ma purtroppo tali emendamenti sono stati "disillusi", perché troppo spesso la burocrazia è più attenta ai calcoli che alle esigenze dei cittadini. Questo lo critichiamo e come Lega difenderemo sempre i nostri cittadini e il nostro territorio *(Applausi)*, perché la Lega è il territorio, è il cittadino,

sensibilità politica, ma un sentimento di appartenenza raro e per questo li ringrazio. Per tornare all'Alitalia, spero che in sede di discussione di bilancio

mia patria - fondatrice dell'Unione europea. Far partire questa compagnia aerea con soli 52 aeromobili è stato un oltraggio alla nostra Nazione. Vorrei ricordare a tutti, soprattutto ora che andremo ad esaminare il disegno di legge di bilancio e successivamente il PNRR, che siamo una penisola e dunque dobbiamo rafforzare il trasporto aereo e il trasporto portuale,

l'abbiamo voluta e la dobbiamo tutelare, affinché non venga fagocitata da altri soggetti o compagnie aeree straniere, anche per tutelare - e qui ribadisco l'importanza del territorio - il turismo italiano. *(Applausi)*. Abbiamo perso tantissimi turisti che vanno in Spagna e in Francia, i cui Governi difendono i loro *asset* principali. Per noi il piano industriale deve essere fondamentale. Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, che hanno presentato un emendamento per tutelare i dipendenti di Air Italy, che sono rimasti scoperti e non hanno garanzia del futuro. Tutti uniti andremo a ripresentare l'emendamento a tutela di questi lavoratori in bilancio. Ora è stato approvato un

dei commercianti esodati, che per un cavillo burocratico - anzi, per una stortura burocratica - non hanno le coperture. Hanno chiuso le loro attività e non hanno la copertura INPS; non hanno la cosiddetta pensioncina. Parliamo veramente di pochissimi euro mensili che, però, cambiano la vita di questi commercianti. Mi riferisco a quei piccoli commercianti, spesso e volentieri attività a conduzione familiare che sono state messe in crisi

forse un po' più personale che di partito, sul reddito di cittadinanza. Vorrei permettermi con la massima umiltà di dare un piccolo contributo alla discussione. Perché non ragioniamo su un accordo Governo-Regioni-Comuni per trasformare il reddito di cittadinanza in borse lavoro per le persone con necessità di lavorare? lavori socialmente utili. In tal modo rimettiamo al centro la persona, le diamo dignità e non semplicemente assistenza, come spesso e volentieri capita con il reddito di cittadinanza. *(Applausi).* Mettiamo al centro la persona, facciamola lavorare. Le persone hanno bisogno di dignità. Abbiamo approvato il famoso decreto-legge dignità? Diamo loro questa dignità, ragioniamoci; la mia non è una provocazione. In qualità di presidente della commissione servizi sociali del Comune di Fiumicino, quando fui consigliere comunale nel mio bellissimo Comune feci questa proposta e funzionò: le persone partirono con contratti a tempo determinato all'interno delle cooperative e spesso e volentieri sono state assunte a tempo indeterminato e oggi svolgono una vita socialmente attiva e inclusiva.

vorrei riallacciarmi alle considerazioni del senatore De Vecchis, che vedo impegnato. Ha detto una cosa interessante anche dai banchi della Lega. considerazioni al ragionamento che noi di Fratelli d'Italia facciamo quotidianamente, e che anche questa mattina mi appresto a rilanciare nel mio piccolo, e cioè che questo Governo di migliori, al netto della grancassa mediatica di cui dispone, al netto della corsa all'applauso ad ogni costo dei giornaloni di regime, di fatto non ha dato vita a provvedimenti che incidano realmente sulla vita dei cittadini e delle imprese. Forse l'unico provvedimento che ha cambiato la vita degli italiani è stato proprio, come diceva il senatore della Lega, il reddito di cittadinanza, che noi, però, a differenza loro, combattiamo. È uno strumento che consente a un ragazzo di vent'anni pieno di forze di percepire 700 euro al mese, quindi disincentivandolo al lavoro, al lavoro, e fa finta di non vedere il diversamente abile, costretto ancora a poco meno di 300 euro, che magari vorrebbe lavorare, penalizzando quest'ultimo nell'ingresso nel mondo del lavoro e facendo finta che non esista. Al netto di questo, i provvedimenti sono stati davvero evasivi e inconcludenti,

una patente per la guida dei camion pesanti costa dai 2.500 ai 3.300 euro, per conseguirla occorrono sei o sette mesi, pensate. Tutto, chiaramente, per arrivare ad avere, in tanti casi, uno stipendio che non supera quasi mai i 30.000 euro annui. In Inghilterra, la stessa identica certificazione si prende in due mesi e costa 300 euro. Questo è il meccanismo, in un mondo globalizzato, del quale facciamo finta di non interessarci. In Spagna, costa 800 euro, in Romania poche centinaia di euro e dopo un mese si ha la patente di guida.

lavoratori stranieri, in particolare dell'Est Europa, perché, come abbiamo detto, lì è più facile prendere la patente, e i costi elevati innescano un meccanismo che disincentiva l'entrata in questo settore da parte di tanti giovani italiani, determinando una gravissima mancanza di

ha stanziato un *bonus* di 1.000 euro per i giovani fino a 35 anni e un rimborso per chi già percepisce il reddito di cittadinanza, ma la cosa incredibile è che lo ha fatto solo per l'autotrasporto di merci per conto terzi, lasciando fuori tutte le altre tipologie di autotrasportatori che così non possono ricevere alcun *bonus*.

alla crescita del settore e che può davvero porsi come una soluzione alla mancanza di autisti, solo che non ci avete dato ascolto, quindi la nostra proposta di estenderlo a tutte le tipologie di autotrasportatori non è stata presa in considerazione. Lo abbiamo chiesto per i bus turistici, l'abbiamo chiesto per gli autotrasporti di ogni settore, ma ancora una volta - e non capiamo il perché - i nostri emendamenti, in particolare un paio, di buonsenso sono stati,

ci ritroviamo ancora una volta a doverci interfacciare con le categorie e con i sindacati portando zero risposte, non capendo perché questo Governo continui ad insistere senza ascoltare chi vuole invece fare qualcosa di concreto per l'Italia e il risultato sarà che si perderanno ancora una volta migliaia di posti di lavoro.

prima di svolgere il mio intervento, vorrei fare una considerazione di carattere generale. Sappiamo che la nostra non è una maggioranza omogenea, che quello attuale è un Governo di unità nazionale.

trovare la sintesi laddove due Presidenti sono del centrosinistra, in particolare uno del PD e uno del MoVimento 5 Stelle, e i relatori ugualmente sono uno del PD e uno del MoVimento 5 Stelle. Senza nulla togliere al lavoro che hanno fatto, politicamente è difficile trattare determinati argomenti e trovare un equilibrio nella soluzione. Questo lo dico a lei, affinché lo riferisca alla nostra Presidente, che agisca in maniera tale che nelle Commissioni, quando si esaminano argomenti di interesse globale, possa essere rappresentata, quanto più possibile, la maggioranza stessa. Altrimenti si arriva a momenti di frizione - per carità, non cercati - su argomenti che dovrebbero invece trovare una sintesi importante ancora prima di essere trattati nella Commissione stessa. Non mi soffermerò su discorsi particolari. Lo lascerò fare a chi interverrà per il Gruppo Forza Italia dopo di me, alla senatrice Toffanin, che sicuramente ha seguito mirabilmente

Abbiamo veramente affrontato con grande decisione e forse con troppa imparzialità la soluzione di determinati problemi specifici. Abbiamo peraltro dovuto esaminare la manovra molto in fretta; il ricorso alle sedute notturne non è un buon viatico per le manovre, per trovare i giusti equilibri. Lo *stress* esiste, non siamo superuomini, siamo uomini (peraltro, con la mia età, lo posso dire ancora di più), che hanno necessità, quando prendono delle decisioni, di avere i tempi per poter riflettere. *(Applausi)*.

stiamo esaminando, il decreto fiscale, avrà grande incidenza e avrebbe necessitato di tempi superiori. Immagino cosa succederà a breve per il bilancio;

forse più, comunque da diversi lustri, è presente nell'agenda politica del Governo. Ciò che dispiace è che si arriva ad una conclusione ampiamente scontata da tempo; ciò che dispiace ancora di più è che i lavoratori, che devono poter recuperare una loro dignità lavorativa, ancora oggi sono messi nelle condizioni di dover sopravvivere

e senza entrare nel merito delle gestioni (purtroppo è arrivata la liquidazione della società) e chi invece proviene da un'attività privata e si vede spogliato di tutto: questo non è equilibrio, Presidente, non è giustizia sociale. Su questo chiedo veramente l'intervento di tutti i partiti, perché la solidarietà e l'equità vengano dimostrate.

ma non c'erano le figure corrispondenti. Ciò vuol dire che non c'è dialogo tra chi dà lavoro e chi deve riceverlo, non c'è formazione. Il nostro maggiore obiettivo dovrebbe essere quello di incrociare i dati tra il mondo del lavoro e l'offerta di lavoro, senza pensare troppo all'assistenzialismo perpetuo. Chi è in reddito di cittadinanza ed è un cittadino occupabile, ma non ha le caratteristiche rispondenti all'offerta di lavoro da parte dell'impresa, deve essere formato. Si spendono 14 miliardi all'anno in reddito di cittadinanza e provvedimenti per la disoccupazione e solo un miliardo l'anno per la formazione. *(Applausi)*. Il Ministro del lavoro

e deve trovarla anche col mondo politico, verificare se i dispositivi che pone in essere riscuotano gradimento da parte del soggetto politico che è il Parlamento, e non spesso - attuare provvedimenti *spot* che sono fini a se stessi, consumano liquidità, ma non producono alcun effetto. Ritengo che investire sulla formazione, la formazione continua a tutti i livelli,

se siamo parte di questo Governo è per senso di responsabilità nei confronti del popolo italiano che ci ha eletto come suoi rappresentanti. Siamo qui per farci carico delle necessità e delle istanze che provengono dai territori. La pandemia non ha messo soltanto a dura prova la tenuta sanitaria e sociale del Paese, ma ne ha stravolto completamente gli equilibri economici, determinando situazioni di criticità, nuovi poveri, situazioni debitorie insostenibili a cui oggi dobbiamo porre rimedio. In questi mesi complicati, insieme ai colleghi del Gruppo Lega abbiamo raccolto le istanze provenienti dal territorio, le abbiamo tradotte in proposte sempre dettate dal buon senso, a volte anche dall'esigenza di chiarire l'interpretazione di norme difficilmente comprensibili. stante l'esigenza di velocizzare l'*iter* di approvazione, gran parte di queste istanze sono state trasferite in ordini del giorno; confidiamo che verranno tenuti in debita considerazione dal Governo nella sua azione futura e sarà nostra cura rammentarlo. Un tema che ci sta particolarmente a cuore e per il quale ci siamo sempre battuti è quello della rottamazione delle cartelle esattoriali. Abbiamo richiesto la rimodulazione delle scadenze delle rate di rottamazione, la dilazione delle rate restanti, la previsione di una nuova rottamazione per le annualità 2018-2019, con l'estensione della definizione agevolata per le medesime annualità delle entrate regionali e degli enti locali, il prolungamento dei tempi per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento e l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione. Ciò di cui hanno assoluta necessità i cittadini italiani è una concreta pace fiscale poter tirare una riga sul passato per poter ricominciare a vivere dignitosamente nel presente e tornare a credere nel futuro. Non si può chiedere l'impossibile a imprese che hanno visto negli ultimi anni perdite di fatturato incalcolabili, a cittadini che hanno subito e stanno subendo ancora le conseguenze della crisi dovuta all'emergenza Covid, a chi ha perso il lavoro o chi vede le proprie entrate considerevolmente ridotte. Un brocardo latino recita: *ad impossibilia nemo tenetur*, nessuno è tenuto a fare l'impossibile, ed uno Stato non può chiedere l'impossibile ai propri cittadini *(Applausi)*, ma deve metterli nelle condizioni di lavorare e di realizzarsi. È altresì necessario far sentire la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini in difficoltà, soprattutto in un momento delicato come questo, con azioni concrete, mirate e subito attuabili. Inoltre, di fronte a problemi congiunturali come l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, il Governo dovrà sicuramente fare uno sforzo ulteriore al fine di non vanificare la prevista diminuzione del peso fiscale. Nell'anno corrente stiamo infatti assistendo ad un costo della bolletta dell'energia elettrica triplicato rispetto al 2020, mentre quello del gas è raddoppiato: spese ulteriori che si sommano alle criticità esistenti e a cui siamo chiamati a rispondere con gli strumenti necessari. Non possiamo costringere le persone a scegliere a fine mese se pagare le bollette o fare la spesa. È pertanto prioritario, per aiutare le imprese e le famiglie, aumentare i 2 miliardi di euro già stanziati, che risultano assolutamente insufficienti a contenere i predetti aumenti. Uno Stato deve aiutare le imprese a ripartire, i lavoratori ad essere tutelati, i giovani ad affrontare il futuro con speranza, le categorie fragili ad essere supportate da una politica reale di inclusione sociale. Soltanto così possiamo ripartire davvero e ridare alla nostra economia e al nostro Paese un rilancio effettivo che non dimentichi e non lasci indietro nessuno. Prima di concludere il mio intervento, vorrei dedicare qualche minuto all'emendamento del senatore Salvini, approvato dalle Commissioni, che rifinanzia il fondo per genitori lavoratori separati o divorziati con 10 milioni di euro per l'anno 2022. Si tratta di contributi che ammontano al massimo a 800 euro mensili, pensati in un primo momento per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di continuare ad erogare l'assegno di mantenimento nella misura in cui la loro attività lavorativa sia stata fortemente ridotta o sia addirittura cessata per via dell'emergenza epidemiologica. Da adesso in poi, grazie all'impegno della Lega, tali contributi saranno erogati anche per il mantenimento dei figli minori conviventi, nonché dei figli maggiorenni con disabilità grave. Si tratta di un emendamento su cui il Gruppo Lega si è impegnato fortemente perché consapevole del fatto che la pandemia ha aumentato le difficoltà di tutti, ma soprattutto delle famiglie con i figli minori e di quelle che devono confrontarsi quotidianamente con il tema delle disabilità; grazie a questo emendamento oggi saranno maggiormente tutelate. Uno Stato, prima di essere esattore, ha il dovere di essere equo e di venire incontro alle esigenze e ai problemi reali dei cittadini italiani. Con lo stralcio delle cartelle esattoriali faremo un primo passo fondamentale nella direzione auspicata per aiutare tutte quelle persone che oggi ci chiedono di intervenire e di farlo non tra un mese, non domani, ma oggi.

fin quando ho potuto, un emendamento che ritenevo e ritengo essere strategico. Di cosa stiamo parlando? Intanto, parliamo di una storia a lieto fine, anche se, nella realtà, come si sia arrivati a questo lieto fine è un po' più complesso. Parliamo di un emendamento che implementava i fondi, già stanziati qualche tempo fa, per la ricostruzione di una infrastruttura importante nella provincia di Savona, crollata nel 2018. Cos'è accaduto? È accaduto che il il commissario, il provveditore, incaricato della ricostruzione, nel tempo ha dovuto sostenere alcune spese. Quindi, gli mancava un pezzettino di

fino a quando, appunto, si è manifestata la possibilità di predisporre un emendamento che implementasse questi fondi. Attenzione: i fondi che si erano trovati avevano un percorso chiarissimo. Non erano altro che uno spostamento, una variazione di bilancio, all'interno del capitolo di spesa del Ministero dei trasporti, che toglieva da una parte e metteva dall'altra. Tutto a posto. Tutto perfetto. Cosa è accaduto? È accaduto qualcosa, in in realtà, di politicamente inelegante. Lo dico a lei, signor Presidente, che so avere una sensibilità nei confronti di questo Parlamento, oltre che per il ruolo, anche perché ho avuto modo di vivere con lei alcune attività parlamentari.

senatorino della provincia di Savona, sai cosa c'è? Non importa che tu faccia questo emendamento; non importa che tu ti sia applicato molto, che ti sia battuto e che abbia cercato i fili da tirare per portare a casa questo risultato. Ci pensiamo noi. Facciamo un atto interno amministrativo e, come per magia, implementiamo questi fondi.

Mi sono chiesto: ma perché non l'hai fatto prima, allora? Perché non l'hai fatto due mesi fa? Perché hai lasciato più di 60 famiglie nell'ansia di non vedere costruita la fabbrica dentro cui andavano a lavorare?

sta che il decreto è alla firma del ministro Giovannini. E il lieto fine sta nel fatto che ieri il presidente d'Alfonso ha suggerito un ordine del giorno che impegnasse il Ministro

risolve la situazione di stallo che si è venuta a creare con le nuove norme introdotte nel decreto-legge n. 121 del 2021, approvato da pochissime settimane, a seguito di un emendamento profondamente sbagliato presentato dal Partito Democratico e approvato alla Camera dei deputati. Si tratta di un problema serio, denunciato da più parti, dal mondo dell'autotrasporto e da quello dell'industria, un grido di allarme che solo la Lega - lo sottolineo - ha raccolto e con la presentazione del citato emendamento ha cercato di risolvere. La norma contenuta nel citato decreto era nata forse all'interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con l'intento di tutelare dal peso dei trasporti eccezionali le infrastrutture stradali, molte delle quali in Italia sono precarie, a partire da ponti e cavalcavia, magari prendendo a riferimento il crollo del ponte Morandi, sul quale però - lo sottolineo - i trasporti eccezionali non sono mai transitati, perché erano vietati. una ricetta profondamente sbagliata. Occorre invece un'altra via per tutelare le infrastrutture stradali, ricorrendo cioè alle manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie e agli investimenti, non scaricando su altri il problema realizzando una piattaforma nazionale digitale delle costruzioni nell'ambito del più ampio progetto europeo. La Lega in tal senso ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che auspichiamo

La norma approvata nel citato decreto-legge n. 121 del 2021 non solo avrebbe rallentato lo sviluppo del Paese, così come stava già avvenendo, non solo avrebbe compromesso la realizzazione dei tantissimi progetti di nuove infrastrutture di quelle contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui il nostro Paese sta scommettendo e ha precisi obblighi di spesa e di tempo; la norma avrebbe anche vanificato gli investimenti delle società specializzate di trasporto, mettendo in ginocchio loro e l'intero settore. Infine, quella norma sciagurata avrebbe determinato, per il trasporto dello stesso quantitativo di merci, la circolazione in strada di un numero elevatissimo di mezzi pesanti (si è calcolato circa tre volte tanto): un paradosso, se ci pensate, in tempo di *green deal,* di decarbonizzazione, di transizione ecologica, in cui l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre l'inquinamento e le emissioni di anidride carbonica per conto della mobilità leggera e di quella pesante. Si andava esattamente nel verso opposto. Come Lega siamo felici che la nostra proposta abbia attivato riflessioni all'interno del MIMS, che ha fatto una retromarcia, e discussioni con noi proponenti della Lega e con gli operatori del settore. Alla fine siamo felici che sia stata approvata

previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa con la Conferenza unificata, dunque con le Regioni. Noi della Lega siamo orgogliosi di essere intervenuti, passando ancora una volta dalle parole ai fatti, come sempre afferma Matteo Salvini, nell'interesse di migliaia di imprese, di famiglie e soprattutto per lo sviluppo del Paese. Concludo sottolineando come questo straordinario risultato, dove vince il sistema Paese, è frutto di un grande lavoro di squadra della Lega, non solo di coloro che hanno firmato l'emendamento, ma anche e soprattutto dei nostri colleghi leghisti che l'hanno strenuamente difeso prima in Commissione bilancio e poi nelle Commissioni riunite finanze e lavoro.

ai componenti della Commissione finanze e, se mi è consentito, innanzitutto ai componenti di Forza Italia all'interno della Commissione. Ho visto che hanno lavorato con un approccio davvero di grande sacrificio, addirittura con sedute notturne; cosa che, a mio giudizio, bisognerebbe in qualche misura evitare per il futuro, anche se mi rendo conto che forse è questa

fiscale, il minor appesantimento possibile del carico tributario nei confronti delle persone fisiche e delle aziende. Siamo infatti sempre stati assolutamente convinti che bisogna spogliare di lacci e lacciuoli, non appesantire i nostri liberi professionisti, i nostri lavoratori autonomi, anche i lavoratori dipendenti e soprattutto le nostre aziende. Ci sono aziende che lavorano per i primi otto mesi dell'anno solo per lo Stato e soltanto nei restanti quattro mesi possono lavorare per loro stessi. Questo è ormai divenuto assolutamente un peso ingiusto che non fa andare avanti il Paese.

alcune aziende e, in modo particolare, i loro dipendenti hanno sofferto più di altri la pandemia. È la ragione per la quale i nostri esponenti di Forza Italia hanno chiesto e più volte ribadito il differimento del pagamento. Abbiamo ottenuto soltanto un differimento di nove giorni sulla scadenza del 30 novembre, arrivando al 9 dicembre che rispetto allo spostamento all'anno 2022, come in effetti Forza Italia aveva chiesto, è troppo poco. però evidente che uno sforzo va fatto. Credo che anche le altre forze di maggioranza siano consapevoli che tutto ciò che riguarda il peso tributario di fisco agli italiani deve essere tenuto in primaria considerazione rispetto al resto. Forza Italia si sta battendo anche per l'eliminazione e l'abrogazione dell'IRAP, una tassa ingiusta. Ci siamo occupati di tali questioni nel decreto fiscale, ma ce ne occuperemo ancor di più nella legge di bilancio. Queste sono le nostre impronte digitali, questo è quello che noi vogliamo far sapere agli italiani. paghino meno tasse possibili in questo periodo e che il differimento in avanti delle cartelle esattoriali sia una questione evidente. Prima di di concludere, esprimo parziale soddisfazione per un mio emendamento, sottoscritto anche dalla collega Toffanin, dai colleghi Mallegni e Floris, sulle misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni sportive, dilettantistiche e professionistiche. C'è un enorme settore, quasi invisibile, del mondo dello sport, che è quello dilettantistico, degli sport che non vanno continuamente in TV,

non hanno avuto la possibilità anche solo parzialmente di ristorare le proprie casse. Si chiedeva sostanzialmente il rinvio di tutti i tributi di quest'anno all'anno a venire;

Se lavoriamo, ma non riusciamo a far approvare al Governo un semplicissimo decreto attuativo del genere, come possiamo pretendere che su provvedimenti più importanti si vada avanti, pur legiferando?

che un senatore, un maschio, sia ancora qui a chiedere che, nell'ambito del decreto fiscale, venga promosso il decreto attuativo. Ne va della faccia e della reputazione di noi parlamentari che ci diamo tanto da fare per promulgare delle leggi.

abbiamo viste approvate diverse nostre proposte. Ringrazio i colleghi della 6a e della 11a Commissione per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Ovviamente noi della 5a Commissione abbiamo accompagnato i lavori, cercando di dare il nostro contributo dal punto di vista finanziario su ogni emendamento. Molto è stato fatto e molto di più si poteva fare. In definitiva, è importante ottenere dei risultati e avere ben presenti le questioni che rimangono aperte per possibili soluzioni future. Guardo all'imminente lavoro e alla discussione del disegno di legge di bilancio e rivolgo un appello ai colleghi e al Governo perché si abbia una gestione ordinata, ma soprattutto chiara e limpida. Sicuramente sarà un lavoro gravoso per tutti. Il mio appello è cercare almeno di iniziare con i migliori propositi. In particolare, oggi mi vorrei soffermare su un emendamento a mia prima firma, che ha trovato il consenso delle Commissioni riunite 6a e 11a, in una in una versione che - seppure non sia a mio avviso ottimale - risolve la questione della doppia agevolazione IMU sulla prima casa per i coniugi con residenze diverse.

che appartengono a nuclei familiari costretti, soprattutto per motivi di lavoro, a vivere in Comuni diversi; oltre a sopportare il disagio di essere in Comuni diversi, sono costretti a a non vedersi riconosciuta alcuna esenzione IMU. Questa problematica si è verificata negli ultimi periodi e in conseguenza di una sentenza della Corte di cassazione, contraria addirittura ai coniugi residenti in due diversi immobili nello stesso Comune, che invece hanno mantenuto il diritto a un'esenzione; che hanno comunque due immobili, ma per i quali non possono sussistere giustificazioni di tipo lavorativo. In realtà, l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, con le sue indicazioni, aveva permesso in passato che si ottenesse la doppia esenzione; invece, con la sentenza della Corte di cassazione, si è aperta la problematica. Con l'emendamento 5.0.100 si dà la possibilità di avere l'esenzione su un immobile e di scegliere su quale immobile far ricadere la residenza principale. Certo - come dicevo prima - avrei preferito che si fosse tornati alla precedente interpretazione dell'Agenzia delle entrate, garantendo

Ma almeno per il futuro si è messo ordine con questo piccolo emendamento. Poiché comunque alcuni Comuni si sono affrettati a fare accertamenti, mettendo in difficoltà le famiglie e sanzionando comportamenti perfettamente legittimi in base all'interpretazione ufficiale precedente, mi auguro che ci sia un'ulteriore sensibilità da parte di tutti per far cessare ogni attività di recupero per gli anni passati da parte dei Comuni, in applicazione della buona fede che ha guidato i comportamenti dei contribuenti, poi penalizzati dalla mutevolezza della giurisprudenza.

dopo infinite ore di dibattito in Commissione, confronti più o meno accesi e discussioni nel merito dei diversi provvedimenti che andremo a votare e su cui mi soffermerò tra qualche istante, mi pare doveroso riportare all'Assemblea un fatto politico per nulla irrilevante. colleghi, in questa bizzarra legislatura, che prima o poi dovrà finire, abbiamo visto cambiare nel corso degli anni diversi Governi, supportati da variegate maggioranze. Siamo passati dal Governo Conte I, sostenuto dagli amici della Lega e del MoVimento 5 Stelle, al Governo Conte II, supportato dal e dai sempre presenti pentastellati e, infine, al Governo Draghi, appoggiato da tutte le forze presenti nelle Aule parlamentari, ad eccezione di Fratelli d'Italia, di cui orgogliosamente faccio parte.

e alla collega Drago, che tutta questa eterogenea maggioranza in realtà sta all'opposizione quanto noi. È un dato ineccepibile, infatti, che moltissimi degli emendamenti presentati da chicchessia in Commissione venivano puntualmente cassati per volontà del Governo, con la tanto celata scusa che non ci sono fondi per alcun cambiamento sostanziale alla manovra. A questo punto è lecito domandarsi se c'è un Governo tecnico, che nulla ha a che fare con i partiti che lo appoggiano, oppure se c'è un Governo politico, in cui però i partiti che lo compongono non hanno voce in capitolo. la verità è che in Commissione non è arrivato altro che un pacchetto già costruito in ogni suo dettaglio, in cui noi - utilizzando un parallelismo natalizio, che spero mi venga concesso non abbiamo potuto far altro che decidere, forse, il colore della carta con cui confezionarlo. Ciò che è emerso e che preoccupa è il totale distacco tra le prerogative del Governo al decreto fiscale e le richieste, quasi sempre bocciate, che noi parlamentari abbiamo il dovere di porre, tramite gli emendamenti. Il problema, però, è che siamo noi parlamentari, che viviamo i nostri collegi di riferimento e conosciamo le esigenze del territorio, a sapere quali sono le reali richieste di coloro che subiranno le conseguenze di questo decreto-legge. Invece, con rammarico, abbiamo assistito all'impotenza dei partiti politici davanti all'assillante presenza della burocrazia ministeriale e governativa, capace di contrastare le naturali richieste che il Paese, specialmente in un momento difficile come questo, ci ha fatto pervenire. Tuttavia, onorevoli colleghe e colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammettere che non possiamo non registrare una preoccupante e ferma volontà da parte del Governo di non ascoltare ciò del Gruppo Fratelli d'Italia - e spesso anche degli altri partiti - abbiamo a gran voce richiesto. Per carità, qualcosa di buono, specie rispetto al passato, è stato fatto. Abbiamo perso traccia - grazie a Dio - di ridicoli provvedimenti come il *cash back* che, infaustamente, qualcuno del MoVimento 5 Stelle voleva ancora, con coraggio, riproporre. abbiamo letto della presenza di un rinvio per alcune scadenze fiscali che avrebbero messo in difficoltà molti contribuenti. Ma la verità, colleghe e colleghi, che votiamo oggi in Aula un provvedimento timido, ancora distante dalle esigenze del Paese. Come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto il possibile e tutto ciò che è giusto fare. Abbiamo ottenuto il passaggio di alcuni importanti emendamenti, come quello sostenuto da me e dai colleghi De Bertoldi, Iannone e Drago, per fare in modo che i dirigenti scolastici possano avere uno scudo rispetto alle responsabilità civili, amministrative amministrative e penali che la pandemia potrebbe comportare in ragione della delicata funzione che svolgono. Da tempo sosteniamo, infatti, che queste figure non possono essere lasciate sole e non possono essere perseguite se svolgono bene il loro dovere nell'applicazione delle disposizioni che il Governo adotta spesso in continua contraddizione. Non solo: abbiamo impegnato il Governo a rivedere le rate per la rottamazione delle cartelle fino al 31 dicembre 2022; così come siamo riusciti a far approvare un altro emendamento per facilitare la possibilità che le casse di previdenza dei professionisti svolgano attività di assistenza verso gli iscritti durante le situazioni di calamità o emergenza.

Avremmo voluto - attraverso i lavori della Commissione - poter essere ancora più efficienti e incisivi. Avremmo voluto concretizzare nostre proposte in grado di attuare alcuni sgravi o aiuti fiscali, in grado di supportare aziende e famiglie italiane. Tuttavia, con dispiacere non possiamo non dichiarare che molto altro avremmo voluto e dovuto fare, ma che a causa della situazione sopra descritta non ci è stato possibile attuare. una nuova occasione persa che ricadrà per l'ennesima volta sulle spalle dei cittadini italiani, che tutti noi avremmo dovuto meglio tutelare.

si va a ottenere una serie di risultati importanti, attesi dal mondo delle imprese e anche da tanti cittadini. C'è una mini proroga delle cartelle: nove giorni in più per il pagamento della rottamazione ter, saldo e stralcio; può apparire poco, ma - considerando quanto accaduto e i limiti di tempo e sapendo che si aggiungono anche cinque giorni di tolleranza - si arriva di fatto al 14 del mese come ulteriore tempo per poter pagare le cartelle stesse. C'è poi emendamento importante, proposto dal senatore Misiani e sottoscritto da diversi colleghi del Partito Democratico, che prevede la possibilità di cumulo tra l'assegno di invalidità e il reddito da lavoro. da lavoro. A seguito di una circolare dell'INPS si era creata una condizione di particolare difficoltà e criticità per molte persone con disabilità. Ebbene, grazie a quell'emendamento si va a riportare chiarezza in una situazione diventata oggettivamente difficile. C'è un allungamento di trenta giorni, da centocinquanta a centottanta, dei tempi per saldare le cartelle sospese durante l'emergenza Covid e ci sarà anche più tempo, fino al 16 gennaio del 2022, per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020 che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 settembre o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre, ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia. C'è poi un importante impegno da parte del Governo sul *patent box*: le forze di maggioranza hanno chiesto al Governo di rivedere le novità sul regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di *software* protetti da *copyright* e brevetti industriali, che era stata contestata da più parti, e il Governo si è impegnato - e lo ringraziamo - a riformulare la norma nelle prossime settimane in legge di bilancio. Vorrei però soffermarmi più lungamente sulle disposizioni a favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico: una norma che è stata approvata dalle Commissioni e che porta ad introdurre una novità assoluta nel nostro ordinamento, con misure a favore delle *startup* sociali innovative, cioè di imprese che decidono di operare non tanto per una ricerca di utile, quanto per la finalità di dare lavoro a persone autistiche, le quali normalmente faticherebbero a trovare una collocazione lavorativa. Le misure prevedono sgravi fiscali e contributivi per le imprese che devono assumere persone con autismo nella misura di due terzi di tutto quanto il personale operativo. Gli utili saranno esenti per cinque anni dall'imposta sul reddito e dall'Irap. Inoltre, c'è un incentivo previdenziale per l'imprenditore che potrà quindi scontare del 70 per cento quanto dovuto in termini contributivi per un triennio. C'è un beneficio importante anche per il lavoratore autistico, con i redditi che non saranno oggetto di imponibile imponibile e con il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi. In questo modo, con l'approvazione di questo emendamento, viene di fatto quasi totalmente assorbito il disegno di legge che avevo presentato due anni fa proprio su queste tematiche e finalità, frutto di un'iniziativa che molti colleghi ricorderanno che si tenne qui in Senato nel luglio del 2019, nella quale due realtà che operano con ragazzi autistici, PizzAut e

ho avuto modo di conoscere molte altre realtà che hanno questa vocazione, e cioè l'obiettivo di operare perché persone autistiche possano essere incluse nella società e soprattutto possano avere un diritto al lavoro. Penso alla Banda Rulli Frulli, Inchiostro, che si trova a Soncino; penso ad Equo Food in Sicilia, in Provincia di Caltanissetta; all'Albergo etico ad Asti, ma che opera anche in altre parti d'Italia e all'estero; ai Gigli del Campo, in Provincia di Milano. Sono tutte realtà innovative che nascono dalla volontà di famiglie e genitori di poter fare qualcosa di più per i propri figli, perché dopo la quinta superiore di fatto cessano i servizi da parte dello Stato. L'autismo è una realtà che coinvolge oggi circa 600.000 italiani: una persona ogni 100 è affetta da autismo. Credo che chiunque di noi qui dentro, per i numeri che esistono, conosca persone affette affette da autismo, famiglie con figli autistici. I dati dell'INPS, che sono stati allegati alla relazione tecnica, ci dicono che in Italia ad oggi ci sono circa 7.600 lavoratori autistici: autistici: praticamente poco più dell'uno per cento delle persone affette da autismo oggi hanno diritto al lavoro. Sono circa 3.500 le aziende che offrono posti di lavoro a queste poco più di 7.600 persone. Ebbene, le norme che le Commissioni hanno approvato e che andremo ad approvare in via definitiva in questi giorni, dopo questa discussione, tendono proprio a favorire l'incremento dell'inclusione sociale e lavorativa di persone autistiche. Nei

o comunque a persone con autismo possibilità nuove, attraverso il lavoro che - come ben sappiamo - è innanzitutto dignità. Altre strade potranno essere aperte grazie alle agevolazioni e alle norme che inseriamo nel nostro ordinamento. È un modo diretto per dare un sostegno tangibile e concreto alle persone che vivono una tale dimensione e alle loro famiglie.

la dimensione della musica. Potrei raccontarvi di chi decide di aiutare la propria famiglia con lo stipendio che è stato finalmente conseguito. Ho assistito il 1° maggio all'inaugurazione di «PizzAut», la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici, alla presenza del presidente Alberti Casellati, che voglio ringraziare non solo per quell'appuntamento, ma anche perché la cena di due anni fa, alla sua presenza, ha messo in moto un lavoro importante. È stato emozionante vedere un ragazzo autistico firmare il suo primo contratto di lavoro. Non sono molti - vi ho citato i numeri - i ragazzi, le persone autistiche che possono farlo; con queste norme apriamo una strada nuova. Credo che sia una scelta, una decisione politica di cui tutti quanti dobbiamo essere fieri.

Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, condivido quanto detto dal senatore Comincini. Credo che il decreto fiscale e la legge di bilancio siano gli atti fondamentali di un Governo o di un Parlamento. Occorre una visione politica ampia, di prospettiva, di proposta, di crescita - come si usa dire adesso - direi anche di libertà, di superamento della fase pandemica e - auspichiamo - *post* pandemica, che obiettivamente è ancora difficile. Altro che società sfilacciata, come diceva De Rita! In certi aspetti è una società a brandelli: le amicizie crollano sulla divisione tra sì vax e no vax; l'odio e l'invidia sociale prosperano, purtroppo (assieme a tanto bene, senz'altro); la situazione sanitaria, se non è grave, è comunque molto seria e deve essere seguita, normata e fatta rispettare. Oggi ci sono forme di protesta che stanno travalicando le norme dell'ordine pubblico e anche quelle della convivenza. Penso che sul provvedimento in esame ogni parlamentare, in una maggioranza così larga ma anche eterogenea, possa mantenere una serenità e una piccola differenza di giudizio su alcuni fatti. Mi soccorre l'intuito del presidente Berlusconi che ci sprona ad andare avanti e sprona il Governo Draghi, ma siano ammesse alcune note e alcuni suggerimenti al Governo da parte del Senato.

al contenuto del decreto-legge, dopo le nottate degli emendamenti, in cui più o meno tutti i Gruppi hanno avuto qualcosa, sulla base delle sensibilità diverse e della e della rappresentanza di interessi che a volte non coincidono, ma formano la società italiana: sulle proroghe fiscali penso che si poteva e si dovrebbe in prospettiva non è stato possibile questa volta, perché una proroga di nove giorni non è significativa. Penso che chi non riesce a pagare non lo fa apposta, ma proprio non ce la fa, per motivi legati alla propria attività, alla difficoltà di incassare, alla difficoltà di fare utile. Probabilmente quando si fa una proroga - e bisognava farla nell'epoca Covid e tuttora bisogna pensare che poi le scadenze si raddoppiano, gli importi si raddoppiano. Allora bisogna pensare a piani di rientro a lunga e lunghissima scadenza, che fanno cassa nel medio-lungo periodo per l'erario, ma danno anche più facilità a chi si è trovato in difficoltà. Si potrebbero stornare da qualche voce significativa qualche centinaio di milioni per il ritardo in caso di ulteriore impossibilità a pagare, per esempio dal reddito di cittadinanza, ma poi ripristinarlo in corso d'anno.

nella realtà; sono 70-80 miliardi - è conclamato, ma ci vuole un provvedimento che lo certifichi una volta per tutte - per i quali si incassa attraverso l'Agenzia delle entrate dai 6 agli 8 miliardi; qualche volta si è arrivati a 10, ma con un'attività di spesa e di ingolfamento degli uffici molto pesante. Alcuni importi sono residui attivi nel bilancio e bisogna a tutti i costi incassarli, ma entrano tutti gli anni i nuovi importi, per i quali non basta una rottamazione-*ter* o un "saldo e stralcio". Ci vuole qualcosa in più, ci vuole una società che produce ricchezza. Quanto alla riforma fiscale che verrà, che non c'entra direttamente con il dibattito, ma in qualche modo è tirata in ballo, perché soprattutto i giornali economici vi dedicano degli articoli e nei *talk show* televisivi è oggetto di aspettative e condizionamenti, genera in certi casi pessimismo,

per la quale si prevede la trasformazione in sovrattassa, causerà dei problemi ai Comuni che incasseranno in ritardo, ma soprattutto che si differenziano sulla deliberazione dell'aliquota. Questa è la democrazia: chi applica il minimale, chi il massimale, chi un'aliquota intermedia; sulla base dell'aliquota, su quanto paga il cittadino, c'è il giudizio politico. In questi giorni

al catasto, oggi c'è un giudizio dell'UPB secondo cui è una riforma che va fatta. Probabilmente, se ci pensiamo, è giusto che sia adeguino in modo equo i valori; ma, se non si vuole troppo ed aumentare la tassazione, probabilmente bisogna ridurre le aliquote di IMU e IRPEF. Intanto, purtroppo, assistiamo a un dibattito politico che non avviene in quest'Aula. Lo dico per titoli, tanto perché siamo qui non a scaldare i banchi, come alcuni giornali e come una certa mentalità corrente che si diffonde e che viene alimentata ad arte vorrebbe far credere. È stato stipulato un accordo Italia-Francia di cui non sappiamo i contenuti; è vero che ha delle parti segrete e le deve avere, ma io con la Francia andrei molto cauto. Ci sono dei Ministri che parlano di legalizzazione della cannabis; decidiamolo una volta per tutte: consegniamo la dose annua ai primi dell'anno e non se ne parli più. Abbiamo rischiato di non poter dire "buon Natale" in questi giorni, secondo una disposizione della UE, che peraltro poi ci dice dice che comunque dobbiamo tagliare il debito e le spese. Sono le cose che ci dice da sempre. Il caro energia: bisognerà intervenire in qualche modo per eliminare quel meccanismo perverso, ma trovare dei fondi - e sono miliardi

Abbiamo letto su un importante quotidiano che un senatore a vita ha parlato di sospensione della democrazia e dell'informazione, e non fa neanche più scandalo. Io sono preoccupato di queste cose, rispetto alle quali il discorso economico è importante, ma sul quale possiamo trovare la quadra, possiamo trovarci d'accordo tramite emendamenti e norme, perché vedo uno spirito costruttivo nelle Commissioni. Anche l'opposizione gioca il suo ruolo, ma tutto sommato alla fin fine è disponibile. Io obbedisco al motto che è stato alle fondamenta di Forza Italia: in economia tutto è permesso tranne ciò che è vietato, e non il contrario. Pertanto, quando leggo o sento che, siccome c'è la mafia, non facciamo gli appalti, o li ritardiamo o complichiamo alle norme; oppure, siccome ci sono le frodi, facciamo il decreto antifrodi, penso che i cittadini siano tutti onesti salvo eccezioni, che gli organi preposti possono tranquillamente scoprire in pochi minuti. Lo Stato deve ingenerare una mentalità per cui si fa la crescita con norme univoche e chiare, ottimismo, libertà, semplificazione vera, magari un poco di inflazione.

sono contento per il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni nelle Commissioni 6a e 11a. Sono state giornate impegnative devo ringraziare i membri del Governo che ci hanno sopportato e supportato in quelle ore frenetiche, in particolare i sottosegretari Guerra e Freni, che veramente hanno avuto pazienza, e li ringrazio Ma questo non è normale e non dovrebbe essere la normalità nel nostro modo di lavorare. Credo infatti che tutto quello che è stato dibattuto in quelle giornate frenetiche nelle Commissioni sia servito a migliorare il provvedimento. Noi vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il provvedimento e per dare un servizio al Paese. Siamo ben pagati: già che siamo qui, fateci, per piacere, esprimere. Torniamo, se possibile, a una normalità che oggi non viviamo. Infatti anche nel Governo

torniamo a esercitare appieno il nostro ruolo di parlamentari. Il Governo Draghi è nato per combattere la pandemia e tagliare le tasse. Sulle tasse noi siamo partiti dagli ultimi. La Lega ha sempre avuto le idee chiare su cosa ottenere dal decreto. Dopo che maggioranza e Governo hanno trovato l'intesa al tavolo del MEF sugli 8 miliardi per il calo delle tasse in manovra, ora è urgente abbassare i prezzi delle bollette di luce e gas, magari risparmiando sugli sprechi del reddito di cittadinanza. Oggi il costo dell'energia elettrica in Italia ha toccato livelli *record*, mentre il reddito di cittadinanza, come ha già detto il nostro *leader* Matteo Salvini, abbiamo sbagliato ad approvarlo così com'è. La Lega non si arrampica sugli specchi: sulla carta, il reddito di cittadinanza funzionava con un reinserimento al lavoro, ma i dati di reinserimento sono totalmente fallimentari. Quei 9 miliardi spesi così sono un disincentivo al lavoro e noi in Parlamento lavoriamo per eliminare una parte di quella che noi riteniamo una spesa improduttiva ed un incentivo al lavoro nero, ma ne parliamo dopo. Siamo a metà dell'opera. Siamo contenti per il taglio dell'Irpef e dell'Irap. A Draghi chiediamo maggiore coraggio sulle bollette di luce e gas, per le quali serve trovare subito almeno 3 miliardi di euro. Sempre al *premier*, chiediamo la rottamazione delle cartelle esattoriali; chiediamo di alzare il tetto della *flat tax* da 65.000 a 100.000 euro. Significa aiutare il Paese. Togliere un po' di soldi ai furbetti del reddito di cittadinanza e destinarlo ai lavoratori e agli artigiani è cosa utile e da farsi. Questo è un Governo molto particolare, in cui abbiamo scelto di entrare per motivazioni eccezionali. Stiamo pagando, come partito, per questo, ma per noi il partito viene dopo il Paese. Allora, il bicchiere mezzo pieno è che abbiamo salvato la *flat tax*, il forfettario fino a 65.000 euro del fatturato e c'è la proposta della Lega per alzare a 100.000 euro il tetto di fatturato per il regime forfettario semplificato. Speriamo che questa misura possa trovare spazio nella manovra. Il taglio dell'Irpef va bene. Sull'Irap non tutti erano d'accordo. Ci siamo messi di testa dura e abbiamo portato a casa un miliardo. C'è un'odiosa discriminazione tra i lavoratori autonomi, pubblici e dipendenti. Gli autonomi hanno sofferto di più durante la pandemia. Spero che in Parlamento si trovi lo spazio e la voglia comune, che non c'è stata, di investire su un taglio delle tasse e burocrazia, soprattutto per il lavoro autonomo. C'è poi il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali 2018/2019, che è assolutamente emergenziale, e della riapertura dei termini per la dichiarazione per la cassa integrazione e per le rottamazioni precedenti. Il 30 novembre ha rischiato di essere una giornata da ricovero per i consulenti del lavoro Mentre altri si preoccupano del Quirinale, la Lega si occupa di vita reale. Noi per questo siamo pagati. Noi pensiamo che dal catino dei 9 miliardi destinati, spesso a sproposito, al reddito di cittadinanza, si possa, per esempio, trarre denaro altrimenti destinato ai furbetti, agli evasori, agli irregolari e agli spacciatori con Mercedes. La soluzione non è certo quella di scalare 5 euro al mese in caso di mancata accoglienza di proposta di lavoro. Qui c'è qualche miliardo da raschiare e da destinare ad altre voci di spesa. La priorità per la Lega e per l'Italia, invece di parlare del Quirinale, è il taglio delle tasse, quindi penso alla *flat tax.* A oggi sono 1,9 milioni le partite IVA che godono di questa tassazione agevolata e semplificata, molti giovani e molte donne; bisogna però alzare il fatturato da 65.000 a 100.000 euro. Questo significherebbe aiutare altri milioni di lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani che potrebbero abbandonare il divano e cominciare finalmente a scommettere su sé stessi e a investire sul lavoro. Il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali 2018-2019 è una emergenza. Se qualcuno faticava a pagare le cartelle esattoriali prima del Covid, figuratevi dopo un anno e mezzo di pandemia, di chiusure e di *lockdown*. estendere fino al 2019 saldo, stralcio e rottamazione su tutte le cartelle esattoriali inviate; su questo le risorse si possono e si devono trovare.

Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e non troviamo 50 milioni di euro per aiutare le famiglie che convivono e combattono contro l'autismo.

un'ultima riflessione su questo tema: aumentare di 50 euro le pensioni di invalidità e l'accompagnamento per i disabili che hanno un invalidità compresa tra il 75 e il 99 quindi per i gravi e non per i gravissimi, che sono milioni di donne e di uomini in questo Paese, costerebbe 750 milioni di euro. Pongo all'attenzione del Senato anche questa riflessione: si possono prendere dal *mare magnum* del reddito dei furbetti del reddito di cittadinanza che ogni giorno emergono e affiorano? Il mondo intanto ride di noi, visto che c'è chi viene in Italia una volta al mese per incassare il reddito e poi torna al suo Paese, alla faccia nostra. gli invalidi veri meritino più attenzione e rispetto dei poveri falsi. Non stiamo zitti sul fatto che uno dei grandi costi è quello del caro energia (luce e gas). e gas). A settembre e purtroppo anche a ottobre, fra i 27 Paesi dell'Unione europea, l'Italia ha pagato più di tutti l'energia elettrica: siamo ventisettesimi su 27, primi in questa classifica al contrario. di un carico insostenibile per le famiglie e per le imprese. Il presidente Macron, caro a una parte di questo Parlamento, parlando alla di un Paese con 56 centrali nucleari e sostanzialmente autosufficiente (infatti i cittadini pagano molto meno di noi), ha prospettato un piano per la costruzione di nuove centrali di quarta e ultima generazione a impatto ambientale zero e a scorie zero. Noi siamo circondati nel mondo da 440 centrali nucleari in Stati Uniti, Francia, Slovenia, Finlandia e in diversi altri Paesi e per pura ideologia le contrastiamo, condannando le famiglie a pagare più di tutti gli altri

Noi della Lega non ci stiamo e diciamo chiaro e tondo che faremo di tutto per tutelare il lavoro, il sacrificio e il futuro di centinaia di migliaia di lavoratori del settore balneare, del commercio, degli ambulanti e dei servizi. È una sentenza da quarto mondo.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, trovo doveroso iniziare il mio intervento sottolineando l'importanza sociale che ha avuto il reddito di cittadinanza per il nostro Paese. Molti dimenticano siamo in piena pandemia; quel provvedimento era nato per garantire un'interazione funzionale (veramente funzionale) tra il mercato del lavoro e le imprese, con i centri per l'impiego che non diventassero dei baracconi vuoti, soltanto per garantire un posto di lavoro a degli impiegati pubblici anche volenterosi, ma volevamo realizzare questo sistema. La finalità principale era quella di dare dignità ai nostri concittadini che vivevano o vivono una condizione di svantaggio. Questa si chiama dignità

possa diffondersi tra le forze politiche che hanno puntato un elemento che non tocca il MoVimento 5 Stelle, ma i cittadini. Vi ricordo che toccherete

cosiddetto fiscale andiamo a consolidare il piano di alleggerimento del peso delle cartelle esattoriali già cominciato con il Governo Conte II. Riteniamo infatti che anche per questa via si debba dare un segnale ai contribuenti ancora alle prese con la difficile e progressiva uscita dalla crisi pandemica.

Abbiamo portato prima a fine novembre e, poi, di fatto a metà dicembre, il termine per pagare le rate scadute della rottamazione *ter* e del saldo e stralcio senza perdere i benefici di queste definizioni agevolate. Un passo ulteriore sarà tentato in legge di bilancio. Abbiamo aumentato da 10 a 18 il numero delle rate non pagate prima che scatti la decadenza dei benefici delle rateizzazioni delle cartelle in corso prima della sospensione dovuta al Covid. Abbiamo fatto slittare al 16 dicembre il termine entro il quale vanno pagati gli avvisi bonari, i cui versamenti erano stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Certo, ci sono partite che restano aperte e che dobbiamo finalizzare all'interno della legge di bilancio. Sfruttando l'aumento a centottanta giorni del termine entro il quale pagare le cartelle notificate a partire dal primo settembre, dobbiamo costruire un'altra definizione agevolata. Una rottamazione *quater* che possa guardare ai debiti fiscali relativi al 2018-2019 e che possa guardare anche al 2020. In tal senso il MoVimento 5 Stelle ha presentato emendamenti in tutti i provvedimenti economici presentati nell'ultimo anno e mezzo. In un'ottica di semplificazione e contrasto all'evasione, sempre nella legge di bilancio, come MoVimento 5 Stelle intendiamo portare avanti un meccanismo innovativo di accredito automatico su conto corrente della parte detraibile di alcune spese, *in primis* sanitarie. Si tratta di un meccanismo che avrebbe tanti benefici. Il primo sarebbe la velocità di fruizione della detrazione, senza aspettare i tempi più lunghi delle dichiarazioni dei redditi. Il secondo sarebbe il contrasto ad interessi in chiave antievasione, perché chi spende sarebbe incentivato a usare strumenti di pagamento elettronici e quindi tracciabili. la possibilità di sfoltimento delle famose *tax expenditures* che tanto ingolfano il nostro sistema fiscale. Innovazione e semplificazione sono le chiavi su cui dobbiamo continuare a puntare fortemente per permettere al tessuto economico-produttivo di agganciare la ripresa.

è giusto pagare quel tanto che compete ad ognuno, e lo dico da commercialista oltre che da senatore della Repubblica, affinché il nostro Paese possa ritornare ad essere un punto di riferimento mondiale al pari delle altre potenze mondiali.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

in ordine al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (2426). Il